con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico***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

ai tempi delle guerre tra Israele e Libano, che nei nostri ricordi ci riporta a quasi vent'anni fa, è tornato. Purtroppo nella scorsa notte

La sovranità territoriale - lo abbiamo detto ieri in Conferenza dei Capigruppo - non può essere violata. L'Europa, l'Italia e la comunità internazionale non possono restare a guardare in silenzio. Nonostante la disponibilità del Governo a riferire nelle Commissioni congiunte esteri e difesa di Camera e Senato, noi rinnoviamo, attraverso la Presidenza, l'invito al Governo a riferire immediatamente in Aula, perché questi bombardamenti non possono continuare. Il cessate il fuoco a Gaza e in Libano, per preservare la popolazione, liberare gli ostaggi e riaprire lo spazio della politica, dev'essere un imperativo. Signora Presidente, chiediamo attraverso lei al Presidente del Senato di chiedere al ministro Tajani e al ministro Crosetto di riferire urgentemente al Parlamento italiano. Non possiamo restare in attesa: Israele deve fermarsi bisogna chiamare un *timeout* serio in questo contesto, che è diventato di una gravità inaudita; mentre noi parliamo, perdono la vita civili innocenti, che non c'entrano nulla con questa autentica follia e il Governo italiano non può più restare in silenzio e alzare le spalle. Chiediamo che la

rinnoviamo l'invito fatto ieri in Conferenza dei Capigruppo: speravamo tutti che non accadesse quello che è accaduto questa notte, ma purtroppo è accaduto; il Gruppo Partito Democratico chiede al Governo di riferire urgentemente in Aula.

di utilità anche al Governo parlare in quest'Aula per avere un mandato chiaro da parte del Parlamento al fine di rafforzare l'azione di governo verso una pace possibile nelle terre del Medio Oriente, dove ogni giorno, come ricordava il collega Boccia, muoiono innocenti e persone che non hanno nulla a che fare o a che vedere con i gruppi terroristici, che pure tutti noi riconosciamo essere presenti in quelle aree; l'azione che sta facendo Israele, inconcepibile in questa fase, rischia di portare a un'*escalation* del conflitto, che non vogliamo e non possiamo pensare sia inevitabile. Anche da parte nostra, quindi, c'è la richiesta al Governo di riferire in Aula e non nelle Commissioni parlamentari, perché riteniamo che sia questa la sede dove discutere e confrontarci su un tema così importante e fondamentale per la vita dei cittadini.

si debba fare di tutto per evitare un'*escalation* che sembra purtroppo continuare. Credo che il Governo, la presidente Meloni innanzitutto e il ministro Tajani, anche ieri sera e questa mattina, stiano lavorando proprio in questa direzione, con rapporti ai massimi livelli (tra l'altro, la diplomazia italiana è sempre stata particolarmente efficace e particolarmente ascoltata); ritengo pertanto che ci si debba affidare a questo lavoro

tutti noi possiamo anche avere qualche informazione in più e portare qualche elemento in più. Detto questo, credo che si debba e si possa aspettare l'esito del lavoro in queste Commissioni

divisione anche all'interno di quest'Aula o di quella di Montecitorio. Verifichiamo prima che il lavoro in Commissione possa essere magari più proficuo, come tutti noi - credo - auspichiamo.

francamente non sono preoccupata del clamore che può uscire dal Parlamento; piuttosto, sono preoccupata del fatto che possano essere tenute posizioni in qualche modo divisive, senza un contributo reale al rafforzamento dell'azione diplomatica. Penso che dovremmo cercare, invece, di riportare il più possibile la discussione in quest'Aula. Naturalmente, chi vi parla ha sempre sostenuto che ci fosse un diritto-dovere di Israele di difendersi,

riterremo complessivamente di adottare. Lo spettacolo di una divisione sul tema se sia meglio partire dall'Assemblea o dalle Commissioni, francamente, vista la delicatezza del momento, me lo risparmierei, perché non è nell'interesse della causa, non è nell'interesse della causa, né della preoccupazione che in questo momento legittimamente imprese e cittadini italiani hanno. Signor Presidente, mi rivolgo a lei:

e congiunte, dove qualunque senatore, oltre che naturalmente qualunque componente dell'altro ramo del Parlamento, poteva intervenire e fare domande in modo assai più agile di quanto avvenga in un'Aula parlamentare. Pertanto, il contatto con il Governo c'è ed è del tutto tempestivo, essendo stato programmato prima dell'inizio di questa operazione. La posizione del Governo è peraltro in generale molto chiara. Gli appelli alla

credo che non ci sarebbero ancora elementi. Pur sperando in un evolversi diverso della situazione, l'intervento è assolutamente tempestivo. Domani chiunque potrà partecipare, naturalmente i membri delle Commissioni

Hezbollah è presente ben al di là dei limiti previsti dalla risoluzione delle Nazioni Unite, che negli

centinaia di migliaia di israeliani su una popolazione di otto milioni, non di sessanta milioni (sarebbe come se noi, in Italia, avessimo un milione e mezzo di profughi che non possono vivere nelle loro case, perché bersagliati dal territorio di un altro Stato). Anche di questo bisogna tenere conto. In ogni caso, penso che la Conferenza dei Capigruppo e la Presidenza esamineranno quanto sarà opportuno fare.

Signor Presidente, oggi l'Assemblea esamina un decreto variegato nei contenuti, sicuramente poliedrico, poiché contiene importanti e positive misure a beneficio di lavoratori autonomi, famiglie, imprese ed enti territoriali. Il centrodestra ha sempre portato avanti l'idea che bisognasse intervenire sul fronte fiscale con misure in grado di generare maggiori entrate attraverso norme che non risultassero punitive per i contribuenti, con un fisco amico e attento nei confronti di tanti lavoratori autonomi e partite IVA, che, in passato, si sono trovati ad aprire nel tempo contenziosi con il fisco. Il decreto-legge in esame interviene proprio su questo aspetto, introducendo un'importante novità, dalla quale vorrei partire per analizzare i contenuti del testo e motivare la nostra decisione sul voto finale. Mi riferisco, in particolare, alla nuova spinta impressa dal concordato preventivo biennale, che riguarderà un'ampia platea di autonomi e partite IVA, che potranno aderirvi entro il prossimo 31 ottobre attraverso il ravvedimento speciale. Questa misura, relativa agli anni 2018-2022, per i contribuenti che aderiranno al concordato, appunto preventivo biennale, riguarda una platea di oltre 4,5 milioni di contribuenti, che avranno la possibilità di regolarizzare la propria situazione nei confronti dell'erario a condizioni particolarmente vantaggiose. Si tratta di una misura equa, che permetterà ad un ad un grandissimo numero di partite IVA e autonomi di regolarizzare la posizione con il fisco italiano, con aliquote ridotte, senza sanzioni e in maniera premiante per i contribuenti che nel tempo hanno dimostrato di essere più affidabili. una norma che dimostra una grande attenzione verso la categoria dei lavoratori autonomi, fondamentali per il sistema Paese e che, inoltre, per quanto riguarda gli anni centrali del Covid-19, prevede un'ulteriore diminuzione dell'imposta sostitutiva, proprio a dimostrare quanto dicevamo all'inizio: bisogna andare incontro a lavoratori e imprese che hanno aperto un contenzioso con il fisco per motivi troppo spesso indipendenti dalla loro volontà. Gli autonomi hanno pagato molto caro quegli anni e l'attenzione che dimostra il Governo nei loro confronti attraverso questa misura non fa altro che contribuire a chiudere un periodo complesso, per sostenere e rafforzare ancora di più il rilancio economico che sta vivendo l'Italia. La misura determinerà maggiore gettito a fronte di una riduzione generalizzata della pressione fiscale e, soprattutto, consentirà di incamerare risorse utili per tagliare l'Irpef ai redditi sotto i 60.000 euro. Com'è evidente, il decreto *omnibus* interviene con una misura che non ha effetti solo ed esclusivamente per i lavoratori che ne beneficeranno, ma, a cascata, anche per altre categorie economiche. Pensiamo ora ad un altro capitolo importante, quello che riguarda il PNRR. Grazie all'emendamento contenuto nel provvedimento, il Governo semplifica il processo di erogazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assicurando la liquidità necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti

Questo è un aspetto su cui vorrei focalizzare la parte centrale del mio intervento. L'Italia ha dimostrato di essere il Paese capofila per quanto riguarda il PNRR: con questo Governo siamo stati i primi a ricevere le *tranche* di finanziamento e a presentare i relativi ora dobbiamo e possiamo imprimere un'ulteriore accelerazione con questo correttivo, erogando velocemente le risorse per finanziare il 90 per cento dei costi trasferiti entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta. Andremo così incontro a cittadini ed enti locali che, grazie a queste misure, potranno finalmente beneficiare di opere che modernizzeranno a trecentosessanta gradi il nostro Paese. Quando parliamo di PNRR, parliamo di investimenti che avranno un impatto sul nostro futuro e quindi sulle nuove generazioni. Sono risorse, quelle europee, che vanno messe a terra per il bene dei territori, al di là dei colori di appartenenza. Questo dovrebbe spingerci a fare squadra in Parlamento e, più in generale, a tutti i livelli istituzionali, affinché si raggiunga il traguardo portando a casa tutte le risorse, senza spendere male o in maniera inefficiente neppure un centesimo. Va in questa direzione la misura contenuta nel decreto-legge che approviamo oggi. Si spinge sull'acceleratore per il bene dell'Italia, per il bene e il futuro dei nostri territori. Parliamo ancora di enti locali. Un emendamento approvato ieri nelle Commissioni bilancio e finanze in maniera *bipartisan* estende al 2027 la rinegoziazione dei mutui degli enti locali. Si tratta di una norma che dà respiro a chi ogni giorno si occupa di garantire i servizi ai cittadini delle nostre comunità. Questa misura infatti alleggerisce l'equilibrio corrente degli enti locali, estendendo la possibilità di utilizzare fino al 2027, senza vincoli di destinazione, le economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e prestiti e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dai Comuni. Sempre in tema di enti locali, nelle scorse settimane l'allarme era stato lanciato proprio dall'ANCI: ad oggi, in oltre 2.100 Comuni italiani ci sono soltanto 261 posti di segretari comunali, e questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore.

nell'ottica di superare la cronica carenza di personale. L'emendamento approvato prevede la possibilità di consentire l'utilizzo fino a trentasei mesi di segretari comunali di prima fascia nei Comuni anche per per le amministrazioni non abilitate. Si tratta di una norma importante per rafforzare le amministrazioni e quindi impattare positivamente sulla vita dei cittadini. esame mostra inoltre attenzione verso le famiglie a più basso reddito, in un quadro complessivo di sostegni diretti e indiretti che nel tempo impatteranno positivamente su questa parte della popolazione. Il Governo ha introdotto infatti il *bonus* Natale di 100 euro esentasse, che sarà erogato con la tredicesima mensilità a circa 1,1 milioni di lavoratori dipendenti. Sosteniamo la famiglia e la natalità con il *bonus* che ha un forte impatto sociale, che rafforza il *welfare* familiare e dimostra ancora una volta quanto questa maggioranza e questo Governo siano attenti tanto al mondo produttivo quanto alle fasce più deboli della popolazione, in un'ottica sistemica che non lascia indietro nessuno. Passiamo ora a una misura che va invece a beneficio delle imprese che operano nel settore zootecnico. Vorrei evidenziare lo stanziamento di 10 milioni a chi ha subito i danni causati dalla peste suina, come gli operatori della filiera, e l'emendamento approvato ieri in Commissione sul contenimento dei cinghiali selvatici, per il quale invece sono stati previsti altri 13 milioni: sono due interventi tangibili e concreti, con i quali il centrodestra e il Governo dimostrano ancora una volta attenzione al mondo del settore primario, il mondo agricolo. Questo, onorevoli colleghi, è il nostro linguaggio che ci contraddistingue e ci connota positivamente. L'Italia che produce e che dà lavoro merita la massima fiducia e il massimo sostegno. Questo è lo spirito che ci ha mossi finora nelle azioni intraprese, anche a livello parlamentare, e proseguiremo in questa direzione, convinti che con il sostegno alle imprese l'Italia rinasca, generando posti di lavoro, crescita e sviluppo nei territori. Per tutte queste ragioni, il Gruppo Civici d'Italia-Noi

per me è davvero complicato parlare nel merito di questo provvedimento, perché è semplicemente inammissibile il modo in cui si è lavorato. Non è responsabilità né dei relatori, né dei Presidenti di Commissione:

Ciò significava che i tempi di conversione avrebbero subìto in partenza una contrazione di una ventina di giorni. Quale fretta c'era da parte del Consiglio dei ministri? Se stiamo alle norme contenute, nessuna. Potevano tranquillamente essere emanate nel primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva. Poi siamo andati in Commissione, dove sono stati presentati 700 emendamenti: un numero tutto sommato accettabile per un provvedimento di ordine fiscale e che interviene su tantissime materie. La Commissione poi è scesa attorno ai 400 dopo le dichiarazioni Da lì è stato un continuo rimandare, in attesa di mediazioni politiche maturate tutte in sede extraparlamentare e dei pareri del MEF, che sono giunti solo dopo una lunga attesa e per appena circa 50 emendamenti. Per tutti gli altri, parere contrario e bocciatura, compresi ovviamente quelli del Gruppo per le Autonomie. Gli altri, alcuni molto importanti per le stesse forze della maggioranza, non si possono neppure ripresentare e discutere, perché intanto il Governo ha annunciato il voto di fiducia, l'ennesimo dall'inizio della legislatura. Alla fine della fiera, il contributo del Senato e delle competenti Commissioni si è ridotto, se così si può dire, quasi a una revisione della punteggiatura del testo. La Camera non potrà fare neppure questo: l'imminente scadenza del decreto-legge costringerà i colleghi a una chiacchierata in Commissione e in Aula, per poi votare, anche lì, con la fiducia. Siamo oltre il monocameralismo di fatto, che oramai non scandalizza nessuno e che è diventato la norma per qualsiasi provvedimento che contiene più di tre articoli. Siamo alla spoliazione delle prerogative del Parlamento, ridotto a un guscio vuoto, chiamato a occupare il proprio tempo con iniziative di indubbia creatività legislativa. Abbiamo ormai occupato tutto il calendario con le giornate celebrative che abbiamo introdotto e che andremo ulteriormente a introdurre, oppure moltiplicando le Commissioni parlamentari d'inchiesta, dove - come ha ricordato il Presidente della Repubblica - c'è il rischio di sovrapporsi, se non addirittura a contrapporsi, ad altri poteri dello Stato. La prossima settimana giungerà in quest'Aula il Piano strutturale di bilancio ed è pleonastico evidenziarne l'importanza: sarà il campo da gioco dei prossimi sette anni, con effetti che riguarderanno anche il prossimo Governo. Il Ministro ha già fatto sapere che non potrà essere in Commissione, ma si collegherà da remoto. Insomma, non ci sono neppure le condizioni minime di decoro per un dibattito degno di questo nome. Con questo andazzo non oso immaginare cosa succederà con la legge di bilancio. Se non si è in grado di gestire un numero sostanzialmente limitato di emendamenti, cosa succederà quando se ne presenterà qualche migliaio? La risposta è già nota ed è nell'ordine di scuderia che la Presidente del Consiglio ha già dato alla maggioranza, riportato da alcune testate giornalistiche: non presentate emendamenti. Allora, signor Presidente, non posso che fare un auspicio. Lo faccio con il disincanto di chi sa che questi appelli, anche quando giungono dalle figure apicali delle nostre istituzioni, cadono sistematicamente nel vuoto. nel vuoto. Prendiamoci un impegno tutti, Camera e Senato, a rendere il lavoro delle Commissioni il più agile e corretto possibile, ma il Governo garantisca al Parlamento lo svolgimento delle proprie funzioni. Questo vale anche per il Senato, che esaminerà la prossima manovra in seconda lettura. finanze (MEF) e alla Presidente del Consiglio, che negli anni in cui era all'opposizione è sempre stata una severa fustigatrice delle derive del ruolo del Parlamento. Per tutte queste ragioni, signor Presidente, il Gruppo per le Autonomie voterà contro il provvedimento in

e la terza è che ci si arriva sempre e costantemente con la fiducia. Senatore Lotito, lo dico con grande rispetto nei suoi confronti perché, come ho già avuto modo di dirle in un'altra occasione, lei è il vero capo di questa maggioranza, le porto un enorme rispetto per le battaglie che quasi sempre riesce a condurre, a discapito di questioni

quella che mi sorprende di più in senso negativo nei confronti del Paese è che di fatto, con questo intervento, si dimezzano le risorse che erano necessarie sul tema del rientro dei cervelli. In un Paese che ha il grande dramma della fuga costante di intelligenze e di talenti, che non riescono a trovarvi il luogo giusto per potersi affermare (perché gli stipendi sono troppo bassi, perché la ricerca ha problemi o perché non ci sono condizioni di vita che consentano loro di impegnarsi nel proprio Paese), il fatto di alterare e diminuire gli interventi che, per esempio, il Governo Renzi aveva voluto in favore del rientro dei cervelli è veramente mortificante. Abbiamo visto un ultimo *rush* finale, con la solita propaganda: l'inserimento nella tredicesima mensilità dei famigerati 100 euro.

che la *premier* Meloni faceva quando noi, con l'impostazione degli 80 euro, eravamo arrivati con tutte le mensilità a una grande platea di italiani: all'epoca si diceva che quell'intervento fosse una mancia; ora che l'intervento è esclusivamente per le tredicesime mensilità ed esclusivamente per una certa categoria di ISEE, quindi *una tantum*, non è una mancia. No, quella che cos'è?

Stiamo parlando però di politiche che non sono in grado di risolvere il problema del costo della vita per le persone, soprattutto in un anno in cui, come abbiamo visto, pur nell'ambito di un incremento in termini occupazionali, è aumentato e non è sostenibile per gli italiani.

Intendiamoci, ognuno di questi settori ha una sua dignità e una sua rilevanza. Però, come sarebbe bello

non sei in grado di risolvere il problema dei rifiuti? Hai i rifiuti per strada? Non sei in grado di realizzare un impianto di termovalorizzazione? Allora ti troviamo una soluzione, perché sei il Presidente della Regione Sicilia, dentro questo provvedimento.

in favore della sburocratizzazione, penso che la sburocratizzazione sia un incentivo a favore di chi fa bene. È giusto allentare allentare le procedure, per esempio, come è avvenuto nel cosiddetto decreto Genova, quando si dimostra di saper realizzare un'opera di ripristino del territorio nei tempi giusti. Allora sì che l'eliminazione della burocrazia ha un senso. Se invece si eliminano gare, procedure ad evidenza pubblica e concorrenza in un territorio che invece non dimostra di saper essere all'altezza,

Dovrebbe consistere nella logica per la quale si dà maggiore autonomia ai territori che dimostrano di saper fare di più. Questa è l'autonomia al contrario, oltre che la meritocrazia al contrario.

È un altro tassello della questione. Voi, invece che prevedere un sistema nazionale che dia incentivi e crei meccanismi di lotta alla burocrazia per investimenti complessivi, date una mano, con una logica completamente antitetica alla concorrenza, a un territorio che non è stato capace nemmeno di risolvere l'emergenza idrica in questi anni. Avete inferto un colpo all'università perché il Fondo per la ricerca e la competitività istituito nel 2020 è stato riversato nel Fondo di finanziamento ordinario in modo del tutto illogico. lavorato sul tema dei capitali evasi, drenando le risorse dalla delega fiscale. La famigerata delega fiscale, che doveva rivedere tutto il sistema, pian piano viene asciugata.

veramente una scarsa capacità di rispetto nei confronti delle opposizioni e di chi fa parte di questa Commissione. Infatti, all'ultimo minuto è arrivato, puntuale come la morte, fiscale che rivedeva il prosciugamento in favore del recupero dei capitali evasi. Ora, non è il principio in sé: figuriamoci se siamo contro l'idea che ci possa essere un recupero di capitali da chi in passato non ha fatto bene il proprio dovere ma vuole comunque rimettersi in sintonia con le azioni giuste nei confronti del Paese. Ma a voi sembra normale che la politica in tema fiscale venga ridotta solo ed esclusivamente a questa questione? E che questo avvenga nottetempo, in una seduta della Commissione, Commissione, senza coinvolgimento e rispetto istituzionale da parte della maggioranza? Io penso di no. Insomma, questo decreto-legge non produrrà

propone un'idea di Paese che non è quella che ho in mente io, cioè un Paese che viene premiato se sa fare e non se non sa fare. Ma questo, come dicevo in premessa,

alcuni emendamenti "calibri da novanta", come si usa dire, che hanno allargato di molto l'intervento su una serie di materie. Mi riferisco a due in particolare: uno sul condono fiscale

Questo è il dato. Voi date il "la" al fatto di continuare a non pagare le tasse. E non venite a dirci che sono entrate più tasse, perché stiamo parlando di quelli che le tasse non le hanno pagate; non siete stati in grado di prenderle prima e non le prenderete neanche adesso, con questa impostazione.

che viene dato solo a una piccola platea di lavoratori dipendenti, che però devono avere a

bisogna individuare quel tipo di famiglia e già il fatto di aver adottato un figlio è qualcosa di anormale, perché l'avete specificato nel testo, con dei distinguo inaccettabili da questo punto di vista. Mi sono soffermato su questi due punti, perché sono due emendamenti, uno del Governo e l'altro dei relatori, che sono stati presentati dopo che ci è stato detto che non c'era il tempo, non c'erano le risorse e non c'erano cose da fare. Però si sono trovate le risorse in questa direzione. Allora la domanda è:

non c'è traccia di piano industriale, eppure la produzione delle categorie tradizionali del nostro Paese - l'*automotive* e il tessile - sta registrando, da diciotto mesi, un continuo scivolamento in perdita dal punto di vista delle ore lavorate.

come tutti i colleghi intervenuti prima di me, mi unisco al coro dei ringraziamenti per il lavoro che in queste settimane è stato svolto dai Presidenti delle due Commissioni bilancio e finanze, dai due relatori, dai membri delle Commissioni 5a e 6a e dal Governo, che ha seguito passo per passo la conversione di questo decreto.

ma intervengo anche per spiegare l'importanza del nostro voto favorevole oggi su questo provvedimento, che non è solo un provvedimento fiscale, ma contiene tante altre misure importanti per lo sviluppo, per l'economia, per i territori, per gli enti locali, per le Regioni, per le famiglie.

difficoltà, sta lavorando in un momento anche geopolitico particolare per il nostro Paese. Tanti sono i temi importanti

economici, guardando alla realtà del Paese e alle difficoltà e per questo mettiamo in campo delle misure che vanno in quella direzione. Nell'ambito del mio intervento parlerò anche di questo, ma voglio ricordare

della dotazione economica a disposizione per le nostre imprese. Precedentemente, vi erano diverse zone economiche distribuite a macchia di leopardo sul territorio e la richiesta che veniva dai territori era di riperimetrare, cioè di ampliare queste zone. Noi lo facciamo oggi e lo abbiamo fatto in questi anni di Governo con l'ampliamento delle zone economiche speciali. Tutte le Regioni del Sud oggi rientrano in una grande zona economica speciale. Si è trattato di un grande esperimento anche a livello europeo. È chiaro che qualche difficoltà iniziale si è registrata da un punto di vista strutturale dell'organismo stesso, ma posso assicurare che oggi gli uffici lavorano bene. Grazie a questa misura di semplificazione e di sburocratizzazione, finalmente

ne ho avuti tanti. Sul mio territorio ho tante associazioni dilettantistiche che oggi, grazie a questo provvedimento, hanno la possibilità di poter ottenere dei crediti di imposta

dei *feedback* positivi perché è una norma che va in una direzione importante per poter continuare oggi a stimolare lo sviluppo di queste associazioni.

non dico quotidianamente - delle emergenze. C'è allora un aumento della dotazione del Fondo emergenze nazionali pari a 150 milioni di euro per il 2024. Abbiamo anche tante altre misure che riguardano

dalle opposizioni che hanno lavorato. Ecco perché non si capisce la contrapposizione quando poi anche le opposizioni stimolano il ragionamento e il confronto con la maggioranza, in particolar modo su temi come quelli relativi agli enti locali. Oggi

Abbiamo introdotto il famoso *bonus* dei 100 euro per una platea di circa un milione di famiglie. Si tratta di una misura importante. Certo, anche noi vogliamo una platea più ampia. La vogliono tutti. Oggi comunque dotiamo un milione di nuclei familiari, soprattutto in un periodo particolare, come quello delle feste natalizie, di un potere d'acquisto maggiore rispetto a quello che avevano. Interveniamo altresì su un'altra iniziativa parlamentare che ha suscitato in queste ore scalpore. Noi stiamo affrontando con determinazione, come non ha fatto mai nessuno negli ultimi cinquanta anni, una grande riforma, che è la riforma fiscale, per dare finalmente ai nostri cittadini un fisco equo. Le tasse le devono pagare tutti, ma ne dobbiamo pagare di meno tutti quanti. Stiamo facendo questa grande rivoluzione e abbiamo studiato all'interno della riforma fiscale il cosiddetto concordato biennale preventivo. Lo Stato si mette cioè d'accordo con le partite IVA, con gli autonomi e i contribuenti per il versamento e per il pagamento delle tasse. In questo decreto, con l'iniziativa parlamentare, avendo ascoltato tutte le categorie e i professionisti, abbiamo pensato anche alla possibilità di uno speciale ravvedimento, per poter oggi portare ulteriore gettito nelle casse dello Stato, con un ravvedimento che riguarda gli anni dal 2018 al 2022. Qui non voglio polemizzare sul retaggio antico di qualche formazione politica di sinistra, che parla ancora di condono e non guarda a qual è oggi la situazione reale del Paese. La gente, i professionisti, le tasse le vogliono pagare, ma oggi vi è anche una difficoltà, dovuta al momento particolare storico del nostro Paese.

puntualmente, sempre e tutti gli anni. Quindi, io respingo al mittente le polemiche sulle parole utilizzate (come condono) per quanto riguarda questo provvedimento, quando, invece,

è anche un ordine del giorno, che in quest'Aula tutto il centrodestra ha votato qualche mese fa, quando il cosiddetto disegno di legge sui diritti d'autore, che veniva dalla Camera, era arrivato blindato. Già all'epoca avevamo chiesto, come centrodestra, di intervenire.

Ce n'è per tutti i gusti, incluso il cinema a quanto pare, salvo aver bocciato un nostro emendamento che prorogava il credito d'imposta per il settore cinematografico. Forse questo vi è sfuggito. Devo dire che questo decreto nasce zoppo fin dall'origine, perché non so se vi siete accorti che abbiamo lavorato a tappe forzate in Commissione, con la continua ombra delle tre settimane di ritardo con cui ci stavamo accingendo ai lavori su questo provvedimento fondamentale per il Paese. il Consiglio dei ministri ha pensato bene di approvarlo, di vararlo, il 9 agosto, quando entrambe le Camere avevano già sospeso i lavori. Evidentemente, i Ministri si erano distratti e non si erano accorti che i loro parlamentari erano già sdraiati al mare, su una bella spiaggia ben attrezzata. Dopo questa piccola distrazione ci siamo accinti con fervore a portare avanti questo provvedimento così mirabolante, come descritto con enfasi dal collega Damiani. Il problema è che

innovativa tanto che ricalca quasi fedelmente l'esperimento fallito vent'anni fa dal vostro ministro Tremonti (quindi, insomma, l'innovazione è proprio il vostro forte); ebbene per chi le tasse non le paga o le vuole pagare il meno possibile o le vuole evadere avete trovato due spiccioli in confronto ai 100 milioni per le famiglie: la finanziate solamente con 990 milioni. Che saranno mai 990 milioni per gli evasori? Questo è il vostro modo di ragionare e di strizzare l'occhio ai furbetti, e lo fate sempre perché evidentemente sono il vostro bersaglio preferito, in senso positivo ovviamente. Abbiamo sentito il senatore Damiani insistere che il ravvedimento non è un condono: una sottigliezza semantica scritta nella norma che però nei fatti si scontra dolorosamente con la realtà.

voi strizzate l'occhio; gli dite che non farete controlli su quello che ha pagato o non pagato tra il 2018 e il 2022; e, siccome questo concordato è proprio indigesto (tant'è vero che l'avete già modificato diverse volte prima ancora che entri in vigore), gli fate pure il ricattino di sottofondo dicendogli che, se non aderirà,

Tutto questo - lo ricordo - alla modica cifra di quasi un miliardo, mentre strizzate l'occhio a chi fa montagne di soldi, come colossi del *web* e banche. Lo sapete che i profitti delle banche italiane sono notevolmente superiori rispetto a quelli delle banche di tutti i Paesi che ci circondano, come Francia e Spagna? La famosa tassa sugli extraprofitti la volete fare, ma non la volete fare; l'avete scritta ma l'avete modificata; adesso siamo al punto in cui la norma sugli extraprofitti diventa un contributo volontario, però, siccome non sapete bene come scrivere il contributo volontario, ve lo state facendo scrivere direttamente dalle banche, tant'è che questi vi hanno rifilato una sola anche stavolta, e invece di un contributo volontario si stanno mettendo d'accordo per un anticipo di liquidità. Perfetto, ci manca solo che poi sui colossi del *web* vi mettiate d'accordo col vostro amico Elon Musk e abbiamo chiuso il cerchio. Una nota a margine, signora Presidente. La Presidente del Consiglio ha fatto giusto in tempo ad invitarlo e a farsi consegnare il premio dall'amico Elon Musk, perché tra qualche settimana approveremo qui il disegno di legge Varchi - spero di no, ma sciaguratamente temo di sì quello che rende reato universale la gestazione per altri. Insomma, ha fatto giusto in tempo a farsi le foto di rito prima che l'amichetto, che ha due figli fatti con la gestazione per altri, diventasse criminale universale *(Applausi)*. Vorrei vedere poi come farà a farsi le foto di rito in futuro. Queste sono solo alcune delle contraddizioni che tanto piacciono alla maggioranza. Passiamo oltre. Che altro c'è in questo mirabolante decreto-legge? Il *bonus* Natale: fate credere con tutti i vostri annunci ai cittadini italiani che date loro 100 euro in più a Natale. Wow, che bravi che siete, peccato che non è niente di nuovo, perché semplicemente state anticipando quello che l'anno scorso, anzi a gennaio, avete chiamato *bonus* Befana. Siccome però avete le elezioni in tre Regioni, avete pensato bene di anticiparlo un pochino, non sia mai che vi dà una spintarella, visti i disastri che avete fatto sul territorio *(Applausi)*. Quello che non dite alle famiglie è che questo non è proprio un *bonus* per tutti, perché è l'emblema di quello che considerate voi il panorama della struttura sociale italiana, perché va alle famiglie monoreddito con coniuge e figlio a carico. Non basta solo il figlio a carico, ci deve essere anche il coniuge; sì, perché la famiglia perfetta è quella dove papà la mattina si alza e va a lavorare, la mamma mette il grembiule, lava i figli, li porta a scuola e poi va a rassettare la casa *(Applausi)*, perché c'è un limite di perché c'è un limite di 28.000 euro di reddito per percepirlo. È a richiesta, tra l'altro, non è nemmeno automatico, quindi questi poveretti lo devono pure chiedere (e se gli sfugge la scadenza, addio *bonus* Babbo Natale, ci vediamo l'anno prossimo). Oltre a doverlo richiedere, se il reddito proviene da un solo componente lo prendono, se arriva da due componenti che guadagnano 12.000 euro l'uno, quindi stanno abbondantemente sotto i 28.000 non lo prendono più. Quindi, mamma cara, devi stare a casa a cucinare: questa è l'idea che avete dell'Italia *(Applausi)*. Lo spiegate benissimo. D'altronde, è di pochi minuti fa un comunicato che ci informa che una consigliera comunale di Forza Italia ha pensato bene di dire che le donne vere sono solo quelle che sono mamme e brave, così dando una bella mazzata tutte quelle donne che, per scelta magari, mamme non lo vogliono essere e sono liberissime di scegliere di non esserlo, e - ancora peggio - a quelle che mamme avrebbero voluto essere, ma non hanno potuto anche per l'idea restrittiva che avete voi della maternità. Con questi 100 milioni potevate veramente fare un favore alle donne e alle mamme, senza stare a guardare reddito, stato civile e compagnia cantando. Potevate quell'IVA che voi avete alzato con la finta scusa che l'abbassamento non aveva prodotto risultati, quando invece i risultati li aveva avuti e sono anche certificati. C'erano state delle distorsioni solo in alcune zone dove c'è poca concorrenza. Ma voi buttate fumo negli occhi. Mi avvio a concludere, signora Presidente, rubando solo qualche secondo in più per dire che

maggiori da parte dello Stato, com'è stato certificato dagli studi che sono stati condotti sugli esiti del *bonus* psicologo. In conclusione, signora Presidente, questo Governo dimostra ancora una volta che non è fatto da incapaci; è solo un Governo neoliberista, austero ed elitario, che strizza l'occhio a chi vuole lui, ai potenti di turno, a una fetta esclusiva della società, oltre che ad amici, parenti, conoscenti e amanti di turno. Mi auguro vivamente che i cittadini italiani si sveglino presto da questa anestesia in cui li avete ridotti, parlando di problemi irreali e irrilevanti, e che lasciate il governo di questo Paese a chi, come il presidente Conte, ha dimostrato con le sue misure di far far girare davvero l'economia, facendo crescere in due anni il PIL del 13 per cento e riducendo il debito del 20 per cento, cosa che voi non sapete fare con una crescita asfittica *(Applausi)*,ancora più bassa di quello che il vostro mirabolante Ministro, che non ne azzecca una in termini di previsioni, aveva preannunciato. Quindi, annuncio orgogliosamente e convintamente il voto contrario del MoVimento 5 Stelle.

non è mai troppo tardi per imparare. Io, per esempio, nel dibattito che si è appena tenuto, e segnatamente nell'intervento che la collega Pirro ha appena fatto, ho scoperto qualcosa della mia gioventù,

Evidentemente, ero in una famiglia riprovevole, che non meritava aiuto. Tuttavia, vi posso assicurare che per l'epoca, per quanto mi ricordo io, se ci fosse stato un Governo che avesse dato un piccolo aiuto a quel tipo di famiglia a basso reddito con papà, mamma e figlio,

o a reddito basso potrebbe anche non essere l'ultimo degli obiettivi per dare un aiuto.

ripetiamo che tanti provvedimenti sono stati approvati in Commissione con il voto favorevole o con l'astensione dell'opposizione e, quindi, evidentemente ci poteva essere un certo

progettare l'automobile nuova: in molti casi quello che ti migliora o ti salva la vita è anche stringere un piccolo bullone. Pertanto, dal nostro punto di vista, questo tipo di

fanno sì che non si paghino né le tasse passate, né quelle future, con il risultato che non ci guadagna oggettivamente nessuno, né il cittadino che non riesce ad avere una vita normale, né lo Stato che non incassa nulla. Pertanto, dal nostro punto di vista, gli strumenti previsti dal decreto-legge in esame sono giusti e voteremo la fiducia. Detto questo, devo però necessariamente sfruttare il tempo che mi viene dato per far capire al Governo che non tutto va benissimo. La definizione stessa di decreto *omnibus* è quella che - secondo me - dovremmo evitare. Capisco che le urgenze ci sono, ma in molti casi

i commissari sono in difficoltà, perché non sono quelli che attengono alla loro area di specializzazione. Io, per esempio, di VPN so abbastanza poco. Una volta ho provato a farlo funzionare perché in aereo non ero consentito usare il mio abbonamento per vedere il calcio. Ma per il resto è ovvio che non sono esattamente un tecnico. Allo stesso modo, su altri aspetti sicuramente all'interno delle Commissioni di merito saprebbero dirmi nel dettaglio le le procedure, mentre si decide di far discutere, per emendamento, qualcosa che non è attinente normalmente alla specificità e alla competenza di una determinata Commissione. doveroso da parte mia richiamare il Governo, per quanto possibile, a garantire *in primis* un'omogeneità della decretazione. Sappiamo che il passaggio successivo, vale a dire

bene, delle istanze che possono essere molto positive non vengono però accettate. Questo lo dico per i tanti miei colleghi

Quanto più i decreti-legge sono ampi come raggio di interesse, tanto più viene il sospetto che ci sia, nella fretta di concluderli e nei tempi stretti per tutti,

è un partito leale che non si tira mai indietro, sempre pronto ad appoggiare e fare squadra, a un certo punto rischia di sentirsi penalizzato perché grida poco su determinati temi o argomenti.

buona parte di tutti questi provvedimenti, soprattutto se ponderati per il valore che impegnano, sono molto positivi per i cittadini e preannuncio Signora Presidente, colleghi, Governo, quando il Governo approva un decreto-legge e lo pubblica l'8 agosto sceglie la strada del non coinvolgimento del Parlamento. Sceglie la strada della confusione. Sceglie la strada della precarietà nel percorso di conversione di un provvedimento, che è stato definito *omnibus*, ma che in realtà affronta questioni corporative, tipiche della destra italiana, che tende a dare risposte individuali di fronte a problemi comunitari. Sceglie la strada della semplificazione, piuttosto che mettersi a lavoro per individuare misure urgenti che sarebbero necessarie e prioritarie per contrastare la precarietà, per aumentare i salari, per garantire diritti di cittadinanza fondamentali quali salute, formazione e istruzione. Senza nulla togliere alle prerogative dei Presidenti delle Commissioni, è stato un percorso tortuoso, determinato da una maggioranza molto confusa, con grandi contraddizioni, che - a nostro avviso - è sempre capace di unirsi sugli obiettivi corporativi (il fisco, ad esempio) e - diciamoci la verità - su misure che hanno inevitabilmente un volto elettorale, anche quando sono sbagliate e precarie.

È una maggioranza che ha mostrato il volto della confusione e della volontà di una lotta interna per occupare il potere. Diciamoci la verità, colleghe senatrici e colleghi un Governo che, di fronte al tema del calcio, su cui in discussione c'è non il merito di un emendamento, ma l'occupazione del potere, la gestione delle federazioni,

C'è sempre la soluzione di problemi corporativi, individuali, utili esclusivamente alla gestione del consenso e inutili a garantire un futuro al Paese. I nostri giovani, Presidente, continueranno a recarsi altrove se non troveranno in questo Paese speranza per un futuro nel quale intraprendere le loro iniziative occupazionali, formative, familiari. Diciamocelo con grande chiarezza: che la destra abbia un volto corporativo a noi è chiaro, lo sappiamo bene. Ma lo vogliamo dire con forza, perché poi sottolineerò sul fisco due questioni molto semplici. Noi abbiamo avanzato - e ringrazio i colleghi del Gruppo Partito Democratico della Commissione programmazione economica, bilancio - proposte alternative, perché abbiamo un'altra visione del Paese, abbiamo altre priorità. Vi abbiamo chiesto di contrastare da subito le discriminazioni, le disuguaglianze, le fragilità, la povertà, le tante solitudini che si ampliano ogni giorno in assenza di interventi urgenti sui salari. Non ve la cavate coi dati sull'occupazione senza andare a guardare cosa c'è dentro quei numeri. Dentro quei numeri c'è precarietà, c'è solitudine, c'è insostenibilità, c'è impraticabilità a costruire la dimensione familiare. Allora come ci rispondete? Ho ascoltato il collega Borghi: arriva il viceministro Leo a raccontarci l'importanza di un *bonus* Befana che va anticipato a Natale. Questa è la grande scelta di questo Governo. E lo fa nonostante le nostre richieste e la nostra disponibilità ad affrontare insieme la modifica dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, che è necessaria. Voi continuate ad avere una visione patriarcale e medievale della famiglia. Non andate da nessuna parte con queste misure, perché ampliano le discriminazioni e creano ulteriori conflitti. Non basta, per le elezioni regionali, dire che si danno 100 euro a un nucleo familiare, che deve avere una moglie e un figlio a carico, senza andare a vedere bene quali sono le priorità e le aree di povertà e di solitudine, senza tener conto del fatto che oggi la famiglia in Italia è plurale. Dobbiamo parlare di famiglie. Dobbiamo parlare di luoghi nei quali la convivenza spesso è necessaria, perché non si hanno le condizioni per investire sul futuro di quel nucleo familiare; quel futuro che voi negate, visto che non state governando per le future generazioni, ma state governando esclusivamente con una visione trimestrale del consenso. *(Applausi)*. Lo dico con grande chiarezza: avete individuato modifiche al concordato preventivo biennale, Presidente, e il meccanismo di ravvedimento consente al contribuente di regolarizzare i mancati versamenti per gli anni dal 2018 al 2022, pagando un'imposta sostitutiva parametrata al punteggio di affidabilità fiscale. Per un mese avete nascosto gli impatti finanziari, agendo con un emendamento del Parlamento.

all'ultima curva, quasi di nascosto e - lo dico, Presidente - dicendo al Paese una cosa vergognosa: usate quasi un miliardo di euro di risorse di finanza pubblica per agevolare l'evasione e l'elusione fiscale, anziché destinarlo ad aiutare le famiglie, a sostenere gli enti territoriali, ad accelerare gli investimenti e a garantire un futuro comunitario a questo Paese.

confondere che questa è una misura che legittima un condono e costa alla finanza pubblica, sottraendo risorse per aiutare le famiglie e le imprese di questo Paese e continuando, Presidente, ad avere un carico insostenibile tutto poggiato sul lavoro e le pensioni. Come faremo a garantire salari più alti, se continuerete a lasciare tutto il peso fiscale sul lavoro e sulle pensioni, ampliando una forbice che compromette

avrebbero voluto annullare l'*iter* penale nel momento in cui si conclude e si completa il debito con l'Erario. quali volete che siano le barriere per pagare le tasse e per non evadere, se addirittura volete eludere il meccanismo che non pagare le tasse è un reato? Vorrei dire con grande chiarezza che tutto questo fortunatamente l'abbiamo fermato, anche attraverso la nostra opposizione e le tante nostre proposte. Avete affrontato il tema della ZES unica, Presidente, sottraendo risorse dal fondo complementare. Avete, cioè, introdotto nella ZES unica meccanismi che non saranno più in grado di andare ad affrontare bene il tema delle aree interne e della riduzione delle disuguaglianze territoriali. E avete cancellato misure che erano previste utilizzando le risorse del fondo complementare, come gli accordi per l'innovazione e la costruzione e il miglioramento penitenziario delle carceri per gli adulti e i minori. Avete sottratto risorse ai piani urbani integrati. Avete, cioè, fatto dei tagli sul futuro del Paese e sulle priorità. E non ho bisogno di aggiungere altro sulle condizioni delle carceri in questo Paese. Tagliate le risorse che nel fondo complementare erano destinate a quegli interventi.

Noi abbiamo scelto di votare contro questo provvedimento perché non garantisce né un futuro alle giovani generazioni, né un investimento sull'impresa e sul lavoro, né una visione di un piano industriale capace di affrontare le transizioni come un'opportunità e non come un peso. Questa sfida non la state affrontando e state lavorando esclusivamente su meccanismi corporativi individuali utili per il consenso, ma negativi per il futuro del Paese.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, voglio innanzitutto ringraziare i Presidenti della 5a e della 6a Commissione, il mio presidente Nicola Calandrini, il presidente Massimo Garavaglia, i colleghi relatori,

oggi in Aula questo documento. Un ringraziamento va anche al sottosegretario Savino, che è sempre stata presente con noi, lo è oggi, ma lo è stata in tutto il corso dei lavori di questi giorni. Si è trattato di andrò poi a definire anche nei suoi contenuti. Ma prima vorrei partire con alcune considerazioni, prima di entrare nel merito, rispetto ad alcune polemiche che ci sono state anche nei giorni scorsi, in particolare quella che faceva riferimento all'uso dei decreti-legge da parte di questo Governo, che sarebbe stato per alcuni eccessivo. per fare un po' di cronaca, mi piace andare a guardare i dati e voglio solo ricordare che il Governo Conte I ha portato a casa 38 decreti-legge, il Conte II ha portati 51, il Governo Draghi ne ha portati 44 e, nonostante la legislatura si sia conclusa prima e quindi abbia avuto un termine inferiore,

Assistiamo poi, in quest'Aula, a un teatrino da parte delle opposizioni, per cui da questa parte la maggioranza sarebbe composta da brutti e da cattivi, da quelli che vogliono in qualche modo soverchiare l'ordine democratico e ridurre il Parlamento a un un giocattolo inutile. Questa è una narrazione che non ci appartiene, ma non lo dico io, lo dicono i fatti, lo dice la storia. In realtà i dati ci dicono che questo Governo ha lavorato bene ed è stato un Governo efficace. I dati ci restituiscono un'inflazione che è assolutamente sotto controllo e non è mai stata così bassa, delle buone *performance* del PIL, dei livelli occupazionali mai così alti.

che è stabile e assolutamente sotto controllo; alla borsa, che procede senza scossoni; alle banche, che sono in grado oggi di sostenere le imprese. Aggiungiamo ancora i dati del PNRR, che mettono l'Italia all'avanguardia rispetto agli altri Paesi europei.

Abbiamo aggiunto 1,6 miliardi agli 1,8 miliardi che erano già stati stanziati: mi sembra un risultato importante, un'attenzione che questo Governo sta dimostrando verso l'area del Mezzogiorno. *(Applausi)*. C'è chi dice che i patrioti stanno dividendo l'Italia e che le risorse sono solo al Nord: questa storia non ci convince e i dati lo dicono, perché vanno assolutamente nella direzione opposta. Ricordo ancora il taglio dei tassi, già annunciato dalla BCE, che apporterà una una spinta significativa all'economia reale. Si tratta di tutta una serie di dati che - fatevene una ragione ancora una volta - ci dice che l'Italia sta bene, che la strada che abbiamo imboccato è sempre meno impervia e la velocità del sistema socioeconomico aumenta. Stiamo, quindi, andando nella direzione giusta.

tutti quegli operatori che, a causa della poca neve, hanno visto comunque ridurre i propri ricavi di oltre il 30 per cento, mi chiedo se si tratta di una mancia *(Applausi)* o forse lo erano i 120 milioni dati

Forse un compendio di alta politica? Credo sia giusto ritornare a quelli che sono i dati reali

che vanno nella direzione opposta rispetto a quella sostenuta da chi ha detto che è una scatola vuota. Non è una scatola vuota, per esempio, la somma di 100 euro *una tantum*, che però verrà data a un milione di lavoratori in attesa che si producano gli effetti del del regime fiscale sulle tredicesime mensilità. C'è poi chi parla di ambientalismo e chi invece fa ambientalismo per velocizzare il completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti in Sicilia, e questo nel solco degli interventi del PNRR e del Piano nazionale complementare. Si prevedono dei maggiori poteri in capo al commissario straordinario. Sono misure che andranno

proceduto esattamente nella direzione che il Governo aveva annunciato e condiviso anche con le minoranze. Abbiamo introdotto le pene fino a un anno di carcere per la pirateria TV sulla trasmissione delle partite di calcio e degli eventi sportivi a pagamento.

avere tentennamenti. Il sistema va difeso e tutelato. Vorrei soffermarmi poi sul ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022, rivolto a quasi 3 milioni di partite IVA che aderiranno al concordato

La norma salva Santa Lucia è stata proposta dai relatori, ma l'abbiamo firmata tutti i membri di Commissione, e tutti l'abbiamo condivisa, perché non potevamo permettere che un presidio di eccellenza come il Santa Lucia

Ecco, allora, un ulteriore atto concreto a sostegno delle realtà della sanità italiana. Aggiungiamo ancora la semplificazione dei processi di erogazione delle risorse del PNRR: sugli atenei, 120 milioni di euro per le attività di ricerca e innovazione in partenariato pubblico privato; il contributo straordinario di 10 milioni di euro in favore degli allevatori colpiti dalla peste suina; ancora, l'accoglimento delle richieste che arrivavano anche dall'ANCI per la riduzione dei tempi per l'immissione dei segretari comunali nei piccoli Comuni. Questa era una norma di buonsenso, che aveva l'obiettivo di calmierare la criticità legata alla carenza dei segretari comunali nelle piccole realtà. Potremmo andare avanti ancora molto, ma credo che ciò sia sufficiente per definire e far capire è un provvedimento con dei contenuti e non una scatola vuota, non un provvedimento che manca di visione. Senza cadere in particolari trionfalismi, bisogna avere il buonsenso di riconoscere che questo Governo ha fatto un grande lavoro in materia economica e fiscale. Le sfide sono sono tante, ma sono finiti anche i tempi degli sprechi e delle mostruosità finanziarie, che hanno messo assolutamente sul lastrico la nostra Nazione, e hanno ipotecato il futuro della nostra Nazione. Noi stiamo facendo un lavoro che fanno i politici buoni, quelli che sono buoni amministratori, esattamente come farebbero i buoni padri e madri di famiglia. Quindi, noi ribadiamo la bontà e la funzionalità di un provvedimento *omnibus* che dà molte risposte e appare come un ulteriore tassello verso la stabilizzazione e la crescita. Per questo, il voto del Gruppo Fratelli d'Italia sarà assolutamente favorevole alla questione di fiducia.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

della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Boccia.

B).* Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 113. La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 16,15, con votazioni alle ore 16,30, così come da accordi tra i Capigruppo.

una nuova finestra"). Comunico che il Parlamento in seduta comune è convocato martedì 8 ottobre 2024, alle ore 12,30, con all'ordine del giorno la votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Signor Presidente, onorevoli senatori, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 1060, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, di cui la 7a Commissione permanente ha concluso l'esame in sede redigente lo scorso 17 settembre. Il disegno di legge, a prima firma dell'onorevole Rizzetto ed altri, era già stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati; nel corso dell'esame in sede redigente, la Commissione ha condiviso le finalità e i contenuti del provvedimento normativo in considerazione dell'importanza di rafforzare la conoscenza della sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei giovani. Si è reso, tuttavia, necessario apportare una modifica di carattere prettamente formale al testo approvato in prima lettura, ciò che comporterà un nuovo passaggio - mi auguro davvero rapidissimo - presso l'altro ramo del Parlamento. L'articolo 1 reca le finalità e l'oggetto del provvedimento. Si tratta di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore. Tali finalità sono raggiunte tramite l'introduzione, operata dal successivo articolo 2, delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. L'articolo 2, costituito da un unico comma, prevede, come appena ricordato, l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica; ciò avviene tramite una novella all'articolo 3, comma 1 della legge n. 92 del 2019 che, nel testo vigente, conferisce al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di definire con proprio decreto tali linee guida, indicando in particolare l'elenco delle tematiche in riferimento alle quali sono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento propri dell'insegnamento dell'educazione civica. L'articolo 2 aggiunge quindi all'elenco di tematiche proprie dell'insegnamento dell'educazione civica le conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. È proprio in relazione a tale novella che si è reso necessario operare la richiamata modifica del testo licenziato dalla Camera. In tale testo la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro era stata aggiunta tramite novella all'articolo 3, comma 1, della legge n. 92, consistente nell'inserimento della lettera Tuttavia, successivamente alla trasmissione del provvedimento approvato in prima lettura, è entrata in vigore altra disposizione che ha richiamato il comma 1, dell'articolo 3 della legge n. al fine di ampliare i contenuti dell'insegnamento dell'educazione civica con la tematica dell'educazione finanziaria. Si tratta dell'articolo 25, comma 1, della legge 5 marzo 2024, n. 21, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali, in vigore dal 27 marzo. Si è reso pertanto necessario correggere il riferimento alla lettera h-*bis* con quello alla lettera h-*ter*. L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria; il suo unico comma prevede che dall'attuazione della presente legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione della stessa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo Come da intesa tra i Gruppi, sospendo la seduta che riprenderà alle 16,30 con il voto degli articoli. *(La seduta, sospesa

Signor Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi, non parlo volentieri, perché si parla di un grande dolore e di una Se vogliamo una non identificazione su questo tema; è come dire che si può morire d'amore.

desiderio d'amore che non si conosce. Morire o ammalarsi di lavoro è quasi la stessa contraddizione. Il diritto-dovere sancito anche dalla Costituzione, ma soprattutto dalla prassi di vita: da quando l'uomo e la donna sono scesi dall'albero e sono usciti dalle caverne, il lavoro ci dà identità, prima ancora che risultati economici. spazio per confrontarsi, ci dà modo di sentirsi persona senza vergognarsi. Purtroppo di di lavoro si muore - e possiamo dare delle cifre - ma, in maniera un po' subdola, ci si ammala

anch'io mi sono impegnato a trovare lavoro. Soprattutto il lavoro, nella mia attività sia sindacale sia di neuropsichiatria, è stato il centro, il fulcro e l'interesse principale della mia vita. Credo, al di là delle note autobiografiche, che il lavoro costituisca le fondamenta profonde e radicate di quella casa meravigliosa, anche se qualche volta di difficile accesso, che si chiama società civile. La consapevolezza che dobbiamo difendere la nostra salute nel lavoro e difendere quella degli altri credo che sia una delle forme più importanti della comunicazione, dell'educazione civica, ma anche del nostro equilibrio mentale. Troppo spesso interessi

che procurano, nel lavoro e nella clandestinità, malattia, sofferenza e morte. Quest'anno - ma le cifre non danno conto, se non in maniera molto magmatica,

che dobbiamo impegnarci tutti a far sì che questo diritto fondamentale non si riduca al minimo a causa del rischio, ma anche che sia la compartecipazione

che qualche millennio fa ci si accordasse, magari tramite grugniti, con una comunicazione non verbale complicata, per lavorare tutti insieme, per abbattere un albero

per farlo meglio e in maniera meno rischiosa. Oggi questa comunicazione è sempre portata all'estremo

si sopraffà l'avversario, ma anche l'amico o l'amica, in una realtà incondivisibile di iperproduttività muscolare,

più remunerativo, sia più umano. Qualche volta, quando si costruiva un mosaico, lo si faceva insieme e a mettere insieme le tesserine si gioiva, non si scansava l'amico o l'amica e spesso le tesserine migliori di un mosaico erano quelle sbreccate, scolpite

perché certamente non voteremo mai contro un tema così importante come quello che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro. Contemporaneamente, non possiamo votare a favore, perché - com'è stato detto anche nel dibattito dei colleghi nell'altro ramo del Parlamento, alla Camera - questo provvedimento purtroppo rischia, ancora una volta, di rimanere una legge manifesto,

Siamo tornati spesso su questi argomenti, anche in altri provvedimenti più specifici, però, se si vuole inserire questo tema così importante del rispetto e della conoscenza, allora bisognava prima di tutto mettere le risorse economiche, per quanto riguarda la formazione di chi poi dovrà parlare di questi argomenti e insegnare ai ragazzi un tema così delicato e complesso. Qui, ancora una volta, non ci sono risorse economiche e soprattutto - noi lo sappiamo bene - si destina soltanto un'ora a settimana all'educazione civica. Allora come Gruppo parlamentare ci interroghiamo anche su questo: se si voleva fare qualcosa di positivo per i nostri studenti, per la conoscenza e l'approfondimento di una materia così complessa, bisognava prima di tutto aumentare le ore di educazione civica. È questo l'appello che noi rivolgiamo

dobbiamo prima di tutto chiederci se ci sono le risorse economiche e chi si dovrà occupare dell'insegnamento nelle scuole

soltanto a questo Governo, ci mancherebbe, perché purtroppo questa è una piaga che ci portiamo da anni. Quando però si decide di intervenire con strumenti che dovrebbero andare nella direzione di migliorare e di investire nella formazione e nella sicurezza, di fronte soltanto (basta leggere l'articolo 3 del provvedimento in votazione) quasi a un ricatto morale. Per tutte queste ragioni, con grande dispiacere, non possiamo esprimere un voto favorevole, mentre, per esempio, avremmo voluto che ai ragazzi fossero insegnati anche gli strumenti di base su significato e conoscenza di rispetto dello Stato, sulle norme costituzionali basilari per andare incontro a tutta una serie di richieste che oggi la società, più di prima, ci chiede. Ci chiede tanta formazione e tanta competenza. Purtroppo, a tutto questo, ancora una volta, non abbiamo trovato nessuna risposta e nessun elemento di concretezza

o di tutto quello che è conoscenza e formazione, perché, se non c'è sapere e non c'è conoscenza, non andremo a formare adulti migliori. Il pensiero, le idee e soprattutto tutto ciò che dev'essere critica (e il pensiero è critica) devono essere necessariamente l'obiettivo che ci dobbiamo porre, prima di tutto come

abbiamo un ruolo politico importante, perché rappresentiamo le istituzioni, dovremmo legiferare in questo senso: meno provvedimenti *spot*, meno leggi manifesto e più attenzione a quello che, invece, serve oggi per dare un'educazione completa e formativa ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, cercando davvero di costruire un *welfare* che abbia come pilastri le famiglie e le scuole. Tuttavia, se non diamo soldi ma continuiamo a delegarle responsabilità per quello che non riusciamo a fare come società, ancora una volta avremo fallito come Stato. Per tutte queste ragioni, il Gruppo Italia Viva si asterrà sul provvedimento in

di ogni scuola di ordine e grado e non solo nelle scuole secondarie, perché molto spesso si arriva alla fine. Ho provato in altre occasioni, quando facevo un altro lavoro, a intervenire nelle scuole nelle ore che vengono utilizzate per spiegare i diritti del lavoro a chi si appresta a entrare nel mondo

dentro le scuole devono trovare, nella loro programmazione, lo spazio anche per questa formazione. Questo è il limite. Facciamo il conto delle materie che

di fare una buona cosa, che però nella pratica è lasciata alla soggettività del o della docente e che quindi difficilmente è in grado di diventare un elemento programmatorio

Signor Presidente, è un bene che anche i ragazzi possano seguire questa discussione. Non possiamo che partire dal messaggio del 12 settembre del Presidente della Repubblica, lanciato in occasione della presentazione della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia: «Le morti e gli incidenti sul lavoro sono una intollerabile offesa per la coscienza collettiva», così diceva il Presidente della Repubblica; «Svolgere un'attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società non può e non deve implicare rischi per l'integrità degli individui. La sicurezza nel lavoro è condizione necessaria per rendere effettivo il diritto fondamentale e inalienabile alla salute, tutelato dalla Costituzione, che non può trovare limiti nella mancanza o nell'inadeguatezza di misure idonee a rendere il lavoro e i luoghi ove esso si svolge sani e privi di pericoli. Non sarà mai sufficiente l'impegno a questo scopo delle istituzioni e delle parti sociali». Siamo ben consapevoli che tutto ciò che faremo non sarà mai sufficiente, ma lo dobbiamo fare. Ecco allora che con questo disegno di legge si intende aggiungere l'insegnamento della sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'ora di educazione civica negli istituti scolastici, rispondendo in parte a questo monito e a questa esortazione. Siamo consapevoli che alle poche ore di educazione civica che seguono i nostri ragazzi a scuola si chiede tantissimo, probabilmente troppo, ma dobbiamo farlo, posto che i temi da insegnare e da porre all'attenzione dei più giovani sono moltissimi. Non dobbiamo mai dimenticare

ed è ciò da cui dobbiamo ripartire per essere consapevoli e coscienti di ciò che trattiamo. Siamo consapevoli che è necessaria una maggiore attenzione ai rischi e alle misure di sicurezza, che devono essere le più appropriate e puntuali. La patente a crediti, che è una novità, crea una selezione tra le aziende che hanno maggiore sensibilità su questi temi; è chiaro però che serve una presenza più capillare dei controlli, altrimenti anche questo strumento rischia di non essere sufficientemente efficace. Serve anche una cultura della sicurezza sul lavoro, che, nelle poche ore di educazione civica, possa accendere una consapevolezza nelle teste dei ragazzi e nelle loro coscienze, anche perché domani saranno loro i lavoratori e i datori di lavoro. lavoro. Accogliamo l'appello del presidente Mattarella alle istituzioni (quindi anche a noi). Nelle Commissioni d'inchiesta e in quelle di merito che trattano il tema del lavoro sicuro facciamo e faremo le nostre proposte per tentare di ridurre quell'elenco di persone morte ogni anno in Italia per il solo fatto di essersi recate al lavoro. Mentre le sanzioni intervengono (purtroppo sempre dopo), è però certamente da incoraggiare la creazione di una coscienza della sicurezza sul lavoro e di un percorso formativo dei ragazzi che comprenda anche questo tema. Questo credo sia nostro compito. Anche per questa ragione e forti di questa sensibilità, confermiamo il voto favorevole dei senatori di Forza Italia a questo disegno di legge.

nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica». Qui si toccano almeno due temi molto importanti, quello dell'educazione civica (quindi il percorso scolastico) e quello enorme della sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda il tema dell'educazione civica, va detto che si parla di un monte ore di

dev'essere organizzata bene perché possa essere efficiente e anche sostenuta dal punto di vista finanziario, per non rendere questo un provvedimento *spot*, con un bel titolo e un bel nome, ma di fatto poi totalmente inefficiente e inefficace rispetto agli obiettivi. Tra l'altro, i temi portanti e i pilastri del tema dell'educazione civica sono assolutamente condivisibili e importanti. Ci sono il tema della Costituzione, quello dello sviluppo economico e della sostenibilità, nonché quello della cittadinanza

che però devono trovare poi una rispondenza nei finanziamenti e nell'organizzazione di quest'ora di educazione civica, il cui principio in assoluto ci troverebbe e ci trova d'accordo.

La grossa mancanza che ha questo testo, quindi, è quella di parlare di cose sicuramente importanti e condivisibili, senza però, dall'altra parte, mettere in campo le risorse per poterle realizzare. Tant'è vero che l'articolo 3 del testo che votiamo oggi recita: «Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica», cioè le scuole devono farsi bastare quei 7 euro. Secondo me faranno un po' fatica. Non si può non parlare, però, oggi, visto il tema che stiamo toccando, della sicurezza sul lavoro, su cui

al giorno; questo vuol dire che nel nostro Paese tre persone la mattina partono per andare a lavorare e la sera non tornano a casa, è un numero drammatico. La tendenza che si registra è negativa: nei primi sei mesi del 2024,

peggiorando. È di questo che vorrei parlare, ossia delle proposte che il MoVimento 5 Stelle fa rispetto a questo tema. Ne vorrei citare principalmente tre. al numero degli ispettori sul lavoro presenti in questo momento in Italia, che sono assolutamente insufficienti e mal retribuiti. Quando ci si pone il tema delle leggi per creare un deterrente rispetto a un problema come quello delle morti sul lavoro, poi bisogna anche porsi quello di chi va a fare i controlli rispetto all'applicazione

e gravissime, che non è semplicemente un testo che chiede di inasprire le pene, ma che prima di tutto lavora sulla prevenzione, che dev'essere il punto di partenza di questo ragionamento. Va ad intervenire, ad esempio, sul decreto-legge n. 81 per chiarire meglio quali sono le responsabilità e le ottemperanze che ricadono sugli imprenditori e per mettere in difficoltà mettere in difficoltà gli imprenditori che, in nome del maggior profitto, mettono a rischio la salute e la vita

perdono la vita sul luogo di lavoro: questo, francamente, è insopportabile. La terza proposta che abbiamo avanzato è quella della Procura nazionale, cioè chiediamo che ci sia un *pool* di magistrati che abbia competenze specifiche rispetto a questi reati per poterli perseguire con maggiore attenzione e per far sì che chi, in nome del profitto, voglia lucrare

drammi come la strage di Brandizzo, le morti sul lavoro di Firenze nel cantiere di Esselunga la tragedia di Luana D'Orazio, a cui noi vorremmo dedicare quel testo di legge. Luana è la ragazza che a ventidue anni ha perso la vita, lasciando un figlio di cinque anni, perché la macchina con la quale stava lavorando non aveva più le protezioni,

Non vogliamo nemmeno più assistere a tragedie come quella di Satnam Singh, il bracciante lasciato morire davanti casa, dopo aver subìto l'infortunio che poi lo ha portato alla morte, non c'è stata nemmeno la pietà umana di prestargli soccorso, ma ci si è preoccupati esclusivamente che nessuno sapesse quello che era successo e così lo si è abbandonato come fosse un oggetto davanti a casa, lasciandolo morire. lasciandolo morire. È chiaro allora che è importante parlare di questo tema all'interno delle scuole, però lo è altrettanto non essere ipocriti e, se si vuole parlare nelle scuole e nei percorsi scolastici, all'interno dell'ora dell'ora di educazione civica, di un tema importante come quello della sicurezza sul lavoro, bisogna anche poi mettere a disposizione delle risorse finanziarie conseguenti, affinché questo progetto sia reale e non semplicemente uno *spot* elettorale. Questo è il motivo per cui il MoVimento 5 Stelle oggi si astiene; condividiamo evidentemente il tema del del documento, ma troviamo che non ci sia alcun riscontro pratico nella mancanza di risorse che questo documento porta con sé. Vorrei dire al Governo che, se vuole fare qualcosa di veramente utile per contrastare le morti sul lavoro, potrebbe leggere il nostro disegno di legge e magari farlo votare.

che ha a che vedere con la prevenzione del rischio e con la costruzione di un equilibrio avanzato, che consenta agli studenti e alle studentesse, ai lavoratori e alle lavoratrici di non sottovalutare i pericoli o le minacce che mettono a rischio la vita delle persone e la sicurezza stessa del lavoro che svolgono. È fondamentale accendere un riflettore e mettere una lente di ingrandimento che permetta di guardare anche da un'altra prospettiva, cioè quella dello Stato che non soltanto legifera, vigila, monitora e sanziona il datore di lavoro, ma cerca anche di offrire ai giovani lavoratori strumenti di conoscenza necessari a comprendere quali sono i propri diritti sul posto di lavoro e i no che

L'auspicio è che si sviluppi un'educazione che promuova una cultura della sicurezza anche nelle aziende, tra i lavoratori e i datori di lavoro. La sicurezza sui luoghi di lavoro dev'essere una priorità in ogni ambiente e la formazione di un tassello fondamentale per rendere il luogo di lavoro stesso sicuro e prevenire così incidenti ed infortuni. Ad oggi, sono obbligatori i corsi di sicurezza sul lavoro per chi è già impiegato. Sono corsi di formazione progettati per fornire conoscenze e competenze ai lavoratori e ai datori di lavoro sulle migliori pratiche per poter prevenire gli infortuni sul luogo di lavoro e la formazione può variare in base alle esigenze specifiche delle aziende o alla natura del lavoro svolto. La moderna concezione di sicurezza sul lavoro che il nostro Paese deve acquistare appieno guarda però a questa disciplina come a un concetto generale, più che a una serie di norme, come una filosofia da perseguire

questo aspetto si porta all'interno di un'offerta formativa, educativa e curriculare e si introduce nell'educazione civica. Voglio ricordare all'Assemblea e ai colleghi che è grazie a un provvedimento della Lega che i nostri ragazzi sono tornati a seguirla nel 2020, con uno stimolo di coscienza comune al bene comune che, inevitabilmente, deve includere la salute e la sicurezza dei lavoratori. Questa formazione si aggiunge a quella obbligatoria, di una durata minima di quattro ore l'anno, già prevista in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro durante i percorsi di orientamento, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008. Abbiamo ritenuto preferibile affidare a un insegnamento trasversale come quello dell'educazione civica l'obiettivo della diffusione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, proprio per centrare la finalità di creare una cultura forte della sicurezza del lavoro e non solo una mera conoscenza del diritto, come se si trattasse solo di nozioni di diritto del lavoro e quindi delle norme vigenti: è un cambiamento epocale, ciò che all'Italia serve di più. L'istruzione ha il compito in primo luogo di trasmettere agli studenti l'importanza di lavorare e di studiare in condizioni salubri. Per loro stessi l'ambiente circostante è una condizione imprescindibile, che che genera benefici dal punto di vista fisico e mentale. Questi insegnamenti devono essere impartiti sin dalla giovane età, perché, se apprendono che non è giusto lavorare in situazioni pericolose e rischiose, saranno poi gli studenti stessi a rifiutarsi di esporsi ad un rischio elevato, consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele degli stessi lavoratori. Mi spiace essere stato costretto a modificare il testo e doverlo quindi inviare alla Camera in terza lettura, ma questo Governo sta lavorando tanto e velocemente, sicché nel testo vi era, purtroppo, un errore formale. Il giorno stesso della trasmissione del testo dalla Camera al Senato è entrata in vigore anche la legge che include l'educazione finanziaria tra i temi da affrontare durante il percorso di educazione civica. Quindi, è stato necessario modificare la lettera di riferimento nell'elenco. Sono certo, però, che gli uffici di entrambi i rami del Parlamento si adopereranno per farci approvare il testo in via definitiva quanto prima. Per questo motivo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito

dal fatto che questo 2024 si sta caratterizzando come un anno drammatico per la sicurezza e per la legalità sul lavoro nel nostro Paese. Un anno che si è aperto con due stragi del lavoro, l'incidente nel cantiere Esselunga di Firenze e l'esplosione della centrale idroelettrica di Suviana sull'Appennino bolognese. Due tragedie che si sommano agli infortuni sul lavoro quotidiani, alle morti che ogni giorno compongono questo drammatico bollettino di guerra, per i numeri sempre crescenti, senza dimenticare la terribile vicenda della morte di Satnam Singh, della quale il collega Pirondini già ha detto. Parlando di cultura della sicurezza, dobbiamo fare ancora di più per contrastare lo sfruttamento del lavoro in Italia, il caporalato, che spesso è nelle mani della criminalità organizzata e delle mafie. Tutto questo non dovrebbe solo indignarci, ma farci assumere ancora maggiore responsabilità come legislatore. I dati INAIL del 2022 ci forniscono una fotografia tragica su questo fronte. Oltre 1.000 vittime e più di 580.000 infortuni. La sicurezza sul lavoro, inutile girarci intorno, è diventata un'emergenza nazionale, ma dobbiamo gestirla con una visione complessa, con interventi sistemici, con risorse finalizzate ad incidere su diversi fronti. Lo abbiamo detto a più riprese durante i lavori parlamentari di questi mesi: la cultura della sicurezza sul lavoro, la tutela della salute nei posti di lavoro, la cultura della legalità e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori deve permeare ogni ambito della nostra società ed essere al centro degli interventi e delle azioni politiche. Questo disegno di legge oggi in discussione poteva fare di più in questa direzione. Non possiamo negare che possa essere un segnale importante portare anche nelle scuole l'insegnamento della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, che questa misura da sola non basta. Non basta per il modo in cui è stata scritta, senza risorse finanziarie aggiuntive, senza il coinvolgimento di chi già oggi svolge un ruolo cruciale per la sicurezza dei lavoratori, le organizzazioni sindacali prima di tutto e le associazioni di tutela. Un disegno di legge scarso di contenuti, che proprio per questo non fa onore al grande tema che intende affrontare. In Commissione abbiamo presentato emendamenti non accolti ed in particolare la proposta di inserire, accanto alla parola sicurezza, la parola salute delle lavoratrici e dei lavoratori e di legalità nel mondo del lavoro. Dobbiamo insegnare anche a scuola che cosa significa legalità nel mondo del lavoro e cosa significa diritti e doveri nel mondo del lavoro. Serve un piano nazionale contro gli infortuni e le morti sul lavoro, una strategia che include anche la promozione, appunto, della cultura della sicurezza, della salute e della legalità. Ci saremmo aspettati un intervento comune e collettivo, perché si tratta di un problema antico e cronicizzato. Voi, invece, avete previsto norme sulla sicurezza per i lavoratori e lavoratrici, prima in un decreto e poi in due collegati dei lavori in discussione, uno alla Camera e l'altro al Senato. Una grande confusione normativa, con il risultato che i passi in avanti sono ben pochi, anche pensando, per esempio, alla gestione degli appalti per le opere edilizie. I dati ci confermano che allargare la catena dei subappalti senza controlli, senza evidenza pubblica, non solo aumenta il rischio di mancata formazione per i lavoratori e le lavoratrici e quindi di incidenti (si veda il caso di Firenze), veda il caso di Firenze), ma rende ancora più complessi i controlli su eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata. In tanti di questi incidenti si è fatto persino fatica a comprendere chi era la ditta subappaltante titolare e responsabile dei cantieri, con una deresponsabilizzazione generalizzata. Bisogna invece partire dall'inizio, dalle premesse. L'unica maniera per affrontare, a nostro avviso, il tema della salute, della legalità e della sicurezza sul lavoro, perché anche di salute si parla nel Testo unico in vigore, è iniziare investendo costantemente e sistematicamente sulla formazione, prevedendo ed impegnando risorse. Serve farlo in maniera precisa, mappando le fragilità e le esigenze delle diverse realtà di lavoro e trovando nuovi modi per uscire dal meccanismo per cui il lavoratore o la lavoratrice, vedendosi proporre lezioni generiche e inadeguate, viva i corsi sulla sicurezza spesso come obblighi inutili. Se faremo questo, mettendo anche le risorse, troverà maggiore significato anche insegnare la cultura della sicurezza, della promozione della cultura della legalità nei luoghi di lavoro e della tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, nelle ore di lezione a scuola. Davanti all'aumento delle tragedie nel lavoro, ci saremmo aspettati un percorso condiviso tra enti, forze sociali e partiti. Non è mai stato accettabile, a maggior ragione non lo è nel 2024, che un cittadino o una cittadina italiana si veda messa nella condizione di dover scegliere fra il proprio lavoro e la propria salute e sicurezza. *(Applausi)*. Entrambi sono diritti sanciti dalla nostra Costituzione e non possiamo più permettere che, per negligenza, carenze di strumenti o fondi, impossibilità logistica o formazione non adeguata, le vite delle persone sul luogo del lavoro siano messe in pericolo quotidianamente. È ovvio che non si possa prescindere dalla scuola come punto di partenza dell'educazione a una cultura della sicurezza, della promozione della legalità e della salute sul lavoro. Per restituirle autorevolezza come entità educante in cui sono applicati i valori democratici del confronto, del dialogo, del riconoscimento reciproco, non sono sufficienti le sanzioni, non sono sufficienti guizzi normativi, lontani dalla realtà delle aule, generici e generalisti. Le ragazze e i ragazzi di questo Paese non sono meri contenitori atti a ricevere acriticamente tutto quello di cui li si riempie, soprattutto se privo di progettualità e visione d'insieme. Lo dico, signora Presidente, perché non possiamo nascondere la durissima bocciatura del Consiglio superiore della pubblica istruzione proprio delle linee guida del ministro Valditara sull'educazione civica. È quasi paradossale ritrovarci in quest'Aula a discutere su una materia così importante dopo i rilievi posti sul documento ministeriale: mancato ancoraggio ai princìpi costituzionali, soprattutto in riferimento alla relazione sociale tra individuo e collettività, sostituita da un approccio individualista. Proviamo a pensare questa critica dentro il dibattito di oggi e come l'assenza di una visione sociale impatti con i principi che volete portare avanti con questo provvedimento. Questo Governo continua ad inserire temi dentro l'educazione civica senza affrontare il tema della formazione, delle risorse per la scuola: un atteggiamento sbagliato e alla lunga controproducente. Ecco perché dico che, se davvero vogliamo parlare di salute, legalità e sicurezza a scuola, parliamo allora dell'adeguamento degli organici e delle retribuzioni, di formazione del personale docente, di dialogo e inclusione, di investimenti in scuole che siano strutturalmente affidabili, funzionali, accoglienti e senza barriere architettoniche. Solo pochi giorni fa è stata discussa in Aula una mia interrogazione che faceva riferimento alla Giornata nazionale per la sicurezza a scuola, un'iniziativa che questo Governo ha di fatto abbandonato da due anni, così come non è stato convocato l'Osservatorio per l'edilizia scolastica. È solo un esempio, ma lascia intendere con chiarezza che non servono delle leggine, buone solo per fare un'intervista; servono interventi strutturali, soprattutto se parliamo di educazione e di sicurezza, della tutela della salute e della legalità sul lavoro. Servono risorse e anche in questo testo non sono state previste, come in tanti altri provvedimenti destinati al mondo dell'educazione. *(Applausi)*. Insomma, serve una chiara volontà politica, la volontà di andare oltre gli *spot*, la propaganda, l'*una tantum*, oltre ai disegni di legge un po' come questo, che gettano molto fumo negli occhi senza offrire nemmeno un barlume di concretezza. Per queste ragioni, signora Presidente e colleghi, a nome del Gruppo del Partito Democratico, dichiaro il nostro voto di astensione sul provvedimento.

ringraziare il sottosegretario Paola Frassinetti per il lavoro che ha seguito sia alla Camera che al Senato. Naturalmente desidero ringraziare la nostra relatrice, la senatrice Giulia Cosenza. Personalmente credo che a questo provvedimento non si possa che esprimere un voto favorevole per il nobile e necessario obiettivo di insegnare, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, le conoscenze di base in materia di sicurezza sul lavoro. Le parole del presidente Mattarella ci spronano a fare di più, ma soprattutto ci dicono che in Italia negli anni scorsi non è stato fatto nulla. A me dispiace sentir parlare di spot, di legge manifesto e di possibilità di votare ben altri provvedimenti, quando nella scorsa legislatura e nei precedenti Governi questi provvedimenti non li abbiamo visti realizzare e non li abbiamo visti approvare. Insomma, non vi abbiamo visto arrivare. Fratelli d'Italia già nella passata legislatura ha sostenuto la necessità di iniziare un lavoro che, partendo dalla prevenzione, non può non prevedere l'affermazione di una nuova cultura della sicurezza. Imprescindibile, quindi, è il ruolo della scuola e pertanto il collega parlamentare Rizzetto, primo firmatario della legge, individua la necessità dell'insegnamento, che in questo testo si concretizza come ulteriore tema di trattazione per l'educazione civica. È chiaro a tutti quanti noi che non basterà questo provvedimento a risolvere il problema, così come non si può però negare l'importanza di puntare anche sulla formazione dei giovani, che saranno i lavoratori di domani e dopodomani. Nella nostra Nazione muoiono tre persone al giorno: molti si ammalano sui luoghi di lavoro e altrettanti rimangono infortunati. Abbiamo un diritto costituzionalmente garantito dall'articolo 32 della nostra Carta, che parla di lavoro in ambiente sano e sicuro. Per conoscere i propri diritti bisogna saper leggere un contratto: è indispensabile, per conoscere condizioni non negoziabili che possano orientare scelte serie di lavoro. Anche valorizzare l'esperienza delle testimonianze dei familiari delle vittime, o di vittime stesse che sono rimaste gravemente lese, rappresenta una concreta occasione di presa di coscienza per gli studenti. Inoltre, voglio ricordare, per chi richiede concretezza e fatti dal Governo, che il Governo è fortemente impegnato e ha già incrementato il Fondo indennizzi per le vittime del lavoro, come sono stati messi in campo ben 900 ispettori in più per i necessari controlli. A questo ritengo importante accompagnare la scelta di questo insegnamento da inserire tra i saperi che formano le nuove generazioni. Pertanto, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia a questo provvedimento. DALLA COMMISSIONE Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione

Signora Presidente, prendo la parola per sollecitare il Governo ad intervenire sulla vertenza Superjet International di Tessera a Venezia, che sta vivendo una forte fase di incertezza per il proprio futuro produttivo e occupazionale. Entro il 31 ottobre prossimo, cioè tra poco tempo, andranno sbloccate le quote azionarie attualmente congelate a seguito delle sanzioni internazionali, dall'attuale azionista russo a un nuovo soggetto che si è proposto. Vi è quindi molta e comprensibile apprensione tra i 115 laboratori e le loro famiglie, che attendono il superamento di questa fase di incertezza e che vorrebbero evitare la chiusura di una produzione così importante. Quella della chiusura sarebbe una ipotesi disastrosa per i lavoratori e per il territorio

strategico e importante per le competenze professionali che ci sono, per l'intero comparto e, naturalmente, per la città di Venezia.

Grazie